Naccarato, sull'incidente occorso ad un elicottero statunitense in provincia di Treviso. Dopo l'informativa del Governo, i Gruppi che lo richiederanno potranno avere cinque minuti per le loro dichiarazioni. Comunico che ho provveduto ieri ad inviare un messaggio all'Ambasciata americana che esprimeva il mio cordoglio personale e quello dell'Aula per le vittime dell'incidente che si è verificato.

sulle nostre *e-mail* e sui nostri siti, oltre che sui giornali. Il grido d'allarme viene dalle associazioni del terzo settore, fortemente preoccupate

e che sono stati accantonati gli emendamenti 4.0.500, 5.130, 5.31 e la votazione dell'articolo 5. Riprendiamo dalla votazione dell'emendamento 8-*bis*.100, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

l'emendamento 8-*bis*.100 cerca di correggere quanto disposto dall'articolo 8-*bis*

Presidente, quando sono intervenuto per illustrare gli emendamenti ho battezzato il testo dell'articolo come tipicamente veltroniano perché è frutto delle *avances*, di una delle tante *avances*, compiute dall'attuale *leader* del Partito Democratico.

retromarce. Su questa linea si espresse Veltroni all'epoca della campagna elettorale per le primarie e a questa linea aderì, per esempio, in maniera esplicita e immediata, l'attuale presidente del Gruppo del Partito Democratico, la senatrice Finocchiaro, ma anche altri illustri ed autorevoli colleghi. E altri colleghi della sinistra - oggi della "Cosa rossa 3" - hanno sostenuto, non da oggi, non da oggi, la necessità di ridurre la compagine ministeriale e di tornare al modello Bassanini. Per queste ragioni l'emendamento presentato dal senatore Calderoli, al quale ho aggiunto la firma ritirando un mio emendamento analogo, mio emendamento analogo, cerca di fare chiarezza. Si vuole o non si vuole che la compagine governativa sia ridotta, che i Sottosegretari siano numericamente funzionali alle attività di Governo, non funzionali alla sistemazione di questo o di quel gruppetto che fa parte della maggioranza di Governo? Vogliamo fare questa scelta, sì o no? L'emendamento pone questa drastica decisione:

Noi ci trovammo nel 2001 con la nuova formazione del Governo a ranghi ridottissimi; ricordo che il centro-sinistra all'epoca approvò la nuova organizzazione del Governo, naturalmente cosa fece? Adottò da subito le norme che facevano più comodo al Governo in carica, come la riforma del Ministero delle finanze con l'organizzazione per agenzie e la nomina di consiglieri di amministrazione, ovviamente di area politica ben definita, ma rinviò alla successiva legislatura - quella nella quale abbiamo governato noi - il nuovo assetto di Governo con una molto drastica riduzione dei Ministeri. Noi accettammo quella riforma, anche se ritenemmo opportuno, per una ragione di sostanza e non di poltrone, ripristinare il Ministero della salute, che era stato cancellato dalla faccia dell'organizzazione ministeriale, e il Ministero delle comunicazioni. Ci fermammo a quello e abbiamo sofferto quasi due anni di difficoltà di Governo proprio perché occorreva ristrutturare l'intera compagine. il centro-sinistra è rientrato al potere, è tornato all'antico e ha fatto di peggio. Noi riteniamo sia arrivato il momento di dare un segnale di serietà, di coerenza e di fedeltà a ciò che si va dicendo sui libri, nelle piazze, nelle interviste, nei *talk show*, nelle comunicazioni ufficiali e ufficiose,

È bene che resti traccia nel Resoconto stenografico di una ricostruzione corretta della dinamica che su questo punto, signor Presidente, ha interessato i lavori dell'Aula, della Commissione bilancio e del Senato

contenuto degli emendamenti che io e il collega Bordon abbiamo presentato al decreto-legge che accompagnava la manovra finanziaria. Presidente, ricorderà come io mi ero permesso addirittura di contestare la dichiarazione di inammissibilità provenuta dalla Commissione e poi confermata dalla Presidenza dell'Aula, proprio perché ritenevo che questa materia, essendo sostanzialmente ordinamentale, avesse diritto d'ingresso più nel decreto-legge che non nella manovra finanziaria. Ad ogni modo, ne ho preso atto.

In quel caso il collega Calderoli ha presentato emendamenti che riproducevano la posizione che originariamente era stata nostra, mia e del collega Bordon, oltre che del collega Villone per la Sinistra Democratica. Il

Questo è il senso della questione che abbiamo oggi dinanzi. Si poneva anche un problema pratico e sostanziale che forse presentava pure alcuni riflessi costituzionali. Era possibile imporre

conseguenza dei due decreti‑legge che avevano in qualche modo annullato gli effetti della legge Bassanini era stato il cosiddetto spacchettamento, il quale, al di là di quello che può sembrare a ognuno di noi, produce degli effetti concreti e sostanziali nel momento in cui i Ministeri con portafoglio vengono divisi. Quindi, in

È una composizione che, obiettivamente, per motivi razionali e di organizzazione, non supera la norma Bassanini, ma in qualche modo rappresenta un atteggiamento dei partiti

ricomporre una maggioranza. Tant'è vero, signor Presidente, che la novità sostanziale rispetto alla legge Bassanini è l'aver posto un tetto. Mentre la Bassanini prevedeva solo un modello organizzativo con 12 Ministri con portafoglio,

un ceto politico che nel momento in cui ragiona di ridurre i costi complessivi e impone dei sacrifici riesce a recuperare questo concetto metabolizzandolo fino al punto di dire: "Cominciamo da me".

c'è il riconoscimento di una precisa considerazione: bisogna creare un Governo più agile e rispondente alle esigenze del Paese, capace di parlare la stessa lingua che parla la gente. Se il linguaggio che noi chiediamo alla nostra gente, al nostro popolo è quello del rigore, il Governo dovrà dimostrare che quel linguaggio lo chiede e lo parla per fare in modo che nel Palazzo e fuori dal Palazzo ci sia la possibilità di continuare ad intenderci. È un recupero di sintonia secondo noi essenziale. In questa logica - e concludo

ma non possiamo nemmeno votarli, perché abbiamo partecipato a quel percorso che ci ha portato a condividere una scelta che per fortuna la nostra maggioranza ha condiviso. Quindi, su quei due emendamenti dichiariamo fin da adesso un voto di astensione.

Non siamo in presenza di un'idea economicistica rispetto ad una declinazione che rimane politica. Dico questo partendo dalla premessa che ritengo che il Governo di cui faccio parte abbia una quantità esagerata di Sottosegretari e anche di Ministri: condivido quindi l'opinione che si dà o che si è data rispetto all'opinione pubblica. Ma l'idea per la quale si debbono decidere nella finanziaria i simboli dei partiti, la struttura e l'organizzazione del Governo ritengo sia anticostituzionale e faccia a cazzotti con il buonsenso che è sempre prevalso nelle Aule parlamentari. Per quanto mi riguarda, poiché non ci sono problemi (non so se parteciperò a prossimi futuri Governi), questo è un problema che attiene alla logica politica. So che una delle difficoltà in questo momento rispetto al Paese è anche il numero esagerato di Ministri e Sottosegretari che abbiamo, ma è una questione politica affrontarispetto al proprio elettorato e alla propria opinione pubblica. E che sarà, quando la volta prossima, in presenza di altre vicende di natura finanziaria, si dirà che si ritorna a 20 o a 50 Ministri del Governo? Questo lo decide la maggioranza che è eletta dal consenso popolare, non può essere una decisione all'interno della finanziaria. A questo si oppone la mia coscienza di parlamentare da tanti anni nelle Aule parlamentari, quindi voterò contro. Capirei e sarei disponibile a votare

per cui - e termino qui con una punta certamente di polemica e di amarezza - un noto *anchorman* ci spiega settimanalmente quello che dobbiamo fare sul piano del rigore e si scopre che guadagna un miliardo e mezzo di lire, mi rifiuto!

a titolo personale, come legittimamente può fare, perché il Governo si è dichiarato favorevole alla proposta - ha espresso considerazioni critiche sull'inserimento nella legge finanziaria della normativa che prevede il ritorno alla legge Bassanini.

perché su iniziativa del Governo si è deciso di inserire in questa materia una serie di misure di cambiamento istituzionale che possano comportare una riduzione dei costi della politica. Non credo sarebbe giusto che ci presentassimo al Paese ristrutturando le comunità montane, piuttosto che l'assetto di governo di Province e Comuni (rispetto ai quali ricordo che si prevede la riduzione del numero degli assessori), mentre, partendo dai rami alti, tutto rimane così com'è. Quindi, la sede è certamente quella propria. Né si tratta di un'iniziativa demagogica, ma di un pezzo di riforma istituzionale - non costituzionale, perché in quel caso la sede sarebbe stata altra di cui il Paese ha bisogno. Non c'è solo lo scandalo del numero crescente e senza paragone dei componenti del Governo, avviato dal Governo Berlusconi e purtroppo confermato dal nostro: c'è anche l'inefficienza profonda e i danni alla competitività del sistema Italia e alla modernizzazione che derivano dalla sovrapposizione e dall'incrocio di competenze e di strutture. Il ministro Bonino - che stimo - segnalava come obiezione alla soluzione che stiamo adottando (ma credo invece che l'indicazione che ne deriva sia nel senso che stiamo procedendo nella giusta direzione) che ancora oggi non si è completata nell'ambito dell'Esecutivo la riorganizzazione delle strutture dipartimentali conseguente al

ho fatto poco fa e che sono preminenti, che dal nostro Governo venga un segnale che - ripeto - non è solo di riduzione - che pure esiste dei costi della politica derivanti dal minor numero di personale di Governo da retribuire, ma anche di riduzione di tutti gli annessi e connessi: segreterie, apparati di consulenza e così via a cascata. Ciò al fine di rendere più efficace l'azione di Governo.

il Parlamento avrebbe presentato, in sede impropria rispetto a quella che la Costituzione prevede per la sfiducia al Governo, una sorta di mozione di sfiducia a tempo. È evidente, infatti, che se si votasse una norma che contenesse l'indicazione di una data precisa e ravvicinata per l'entrata in vigore di questa norma significherebbe un atto di sfiducia preventiva al Governo. Ma la Costituzione prevede, per la mozione di sfiducia, un'apposita normativa e adeguate garanzie perché si tratta di un intervento di grande rilievo. Per questo, non solo voteremo contro gli emendamenti che prevedono un termine all'entrata in vigore della riforma ma, se sarà posto ai voti, voteremo anche contro l'ordine del giorno del senatore Calderoli, esattamente per questa ragione istituzionale. Il senatore Calderoli ha tutte le possibilità di presentare una mozione di sfiducia con la quale, partendo dall'approvazione di questa norma, chiedere al Governo di andarsene, ma non si tratta di un ordine del giorno, tanto meno - mi permetto di dire - "trasversale", perché il problema riguarda il rapporto tra maggioranza e Governo, sia pure sotto forma di ordine del giorno e non di emendamento; tema che non è affrontato con lo strumento proprio. Detto ciò non posso non esimermi, in conclusione, da una considerazione politica. Sinistra Democratica auspica che il presidente del Consiglio, Romano Prodi, utilizzi fin dal mese di gennaio la possibilità che il Parlamento gli offre di dare vita ad un nuovo Esecutivo, snello, rinnovato, con una forte e qualificata presenza femminile di dimensione europea e che, sulla base di una ricontrattazione precisa del programma tra centro e sinistra dell'alleanza, possa affrontare con slancio e determinazione la fase della legislatura che è davanti a noi. Completati i lavori della finanziaria, riteniamo si possa aprire una fase nuova e che l'approvazione di questa norma da parte del Senato

I temi che riguardano l'espressione di moda «costi della politica», anche quando incidono su fatti estranei alla finanziaria, è giusto che stiano in finanziaria. Essi

merita un'osservazione che in privato gli ho già fatto. Noi eravamo anche propensi ieri a stralciare o ad accantonare quella norma, ma debbo cogliere l'occasione - chiederei l'attenzione del Parlamento

perché dobbiamo aspettare? Ci troviamo di fronte ad una intimidazione al Parlamento che avviene a pagamento sul principale quotidiano italiano, dove si diffida il Senato dal votare qualsiasi disciplina sui simboli e si utilizza un simbolo di un Gruppo parlamentare, che non è il mio dell'UDC, e la denominazione di un Gruppo parlamentare che è il mio, dicendo, signor Presidente del Senato, nel suo silenzio innanzi tutto, che noi utilizziamo illecitamente queste denominazioni,

da questo momento noi poniamo una questione politica di una intimidazione al Senato da parte di un Gruppo politico,

alla tesi di uno stralcio e di un accantonamento, chiedo al Parlamento di invertire il nostro ordine dei lavori e cominciare da subito una discussione su un argomento che a questo punto diviene centrale. discutiamo della cittadella democratica, Sagunto viene espugnata. La verità è che diventiamo la casta quando rinunciamo a disciplinare persino le regole in base alle quali arriviamo a sederci qui.

meramente demagogico affrontarlo nella finanziaria, non foss'altro perché il Presidente del Consiglio dichiara costantemente che il suo Governo durerà cinque anni. al nostro esame sia un emendamento che dovrebbe intervenire per impedire o comunque per sanare i costi della politica, ma che entrerebbe in vigore dal prossimo Governo, significa chiaramente che si tratta solo di una presa in giro.

dal nostro punto di vista è un problema culturale. Vede, Presidente, della dilatazione dei costi della politica si è fatto un tema di carattere culturale, con particolare riferimento ad una certa posizione che storicamente in questo Paese ha preso la sinistra. La dilatazione dei costi della politica viene da lontano, cioè dal tentativo di accreditare la necessità di dilatare il livello quantitativo - la sinistra sostiene che sia qualitativo - della democrazia in entrata: quindi, più consigli d'amministrazione, più consigli di istituti, più dislocazione dei centri di potere per impedire la gestione del potere alla vecchia Democrazia Cristiana e ai propri alleati. tesi ingraiana che, come lei sa, è piaciuta anche a De Mita e ad altri sostenitori della democrazia orizzontale. Ora abbiamo sentito il collega Salvi vantare la democrazia tedesca e quella francese; noi potremmo aggiungerci quella inglese (perché no?),

diversamente, ci prendiamo in giro e non ci rendiamo conto che, per esempio, abbiamo due esponenti della sinistra che propongono di ridurre l'indennità dei parlamentari, quando storicamente i parlamentari costano molto e hanno tante prebende per le battaglie fatte, soprattutto, dalla sinistra che candidava i propri funzionari di partito, dopo due legislature li mandava a casa, ma li doveva mettere in condizioni

A titolo personale, peraltro, mi permetto di suggerire agli estensori dell'emendamento

mi permetto di suggerire agli estensori dell'emendamento 8-*bis*.801 - che peraltro approvo - che la materia dell'agricoltura è ormai completamente delegata alle Regioni.

a livello europeo dei Ministri dell'agricoltura che amministra circa il 40 per cento delle finanze comunitarie e, quindi, deve esservi evidentemente una personalità politica e istituzionale con rango di Ministro che partecipi a quel consesso,

un Ministro senza portafoglio alle politiche agricole, alimentari e forestali. Faccio anche presente, Presidente, che a livello comunitario un commissario - in questo caso il commissario Borg - è delegato al coordinamento delle politiche del mare. Credo che, nell'ambito di questo Ministero senza portafoglio per le politiche agricole, alimentari e forestali, dovrebbe essere previsto anche il coordinamento delle politiche marittime, in modo da potersi interfacciare in modo consono con il Commissario delegato a livello europeo.

relativamente ai contenuti dell'articolo 94 della Costituzione che avrebbero reso difficilmente applicabile una norma ordinaria rispetto ad un Governo che ha ricevuto la fiducia delle due Camere,

fare in modo che nel giro di quattro mesi, fermo restando il numero dei Ministri, il Governo pervenga ad un ridimensionamento del numero dei Sottosegretari. Abbiamo fissato un numero complessivo di membri dell'Esecutivo: se

Il secondo tende ad introdurre un termine di efficacia della norma che abbiamo espunto in Commissione. Il terzo, quello presentato dal senatore Calderoli, una sollecitazione, un invito, non ha in sé un grandissimo valore contenutistico; però, il parere è ugualmente contrario perché mi sembra che la norma che fissa per il prossimo Governo l'operatività

Ho ascoltato doverosamente l'allarmato intervento del senatore Rotondi e l'appello che egli ha rivolto a lei per quella che egli ha giudicato una intimidazione nei confronti del Parlamento. Mi sono incuriosito ed ho letto la pubblicità riportata sul "Corriere della Sera", esattamente come ha rivendicato lei di poter fare perché è stata pubblicata questa mattina. Rotondi ha parlato di intimidazione a nome dei due senatori iscritti al suo partito. Presidente, poiché le è stata chiesta un'opinione lei è rappresentativo dell'Assemblea - anche a nome dei tre senatori eletti nel mio movimento, mi preme dirle che anch'io considero un'intimidazione quello che è successo, ma non fatta dalle pagine del «Corriere della Sera», bensì da chi, notte tempo, ha approvato questa norma vergognosa. Su questo le assicuro che ci faremo sentire in Aula, laddove si dovesse provare ad andare incontro alle esigenze di chi vuole impedire che la democrazia sia rappresentativa anche delle forze politiche.

Presidente, il collega Barbato ha colto perfettamente il senso dell'ordine del giorno. È stata fatta una cosa: credo che il Governo debba prendere atto e non sia impegnato in nulla se non a corrispondere

*(Ulivo)*. Signor Presidente, questa mattina il collega Manzione ha esattamente illustrato la posizione del Gruppo dell'Ulivo e indirettamente la posizione dei colleghi del centrosinistra. Esiste una valutazione tutta legata alla norma ed esiste una valutazione ovviamente tutta politica. Ora, la valutazione tutta legata alla norma il Parlamento l'ha più volte fatta, perché ha approvato una legge nella quale era prevista la riduzione del numero dei Ministri. Con l'articolo che ci accingiamo ad approvare oggi, in fondo, si ripristina una norma esistente. C'è poi una valutazione politica, la valutazione politica che abbiamo fatto è quella di applicare questa norma con il Governo successivo a quello attualmente in carica. politica la maggioranza ha trovato un suo punto di equilibrio. È evidente, Presidente, che una norma votata dal Parlamento ha un peso

Presidente, alla luce della riformulazione del dispositivo, ritengo doveroso modificare il parere espresso, nel senso di esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno, anche alla luce delle considerazioni

MANZIONE *(Ulivo)*. Signor Presidente, se l'ordine del giorno è trasformato così come lei ha comunicato all'Aula, è un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a valutare il comportamento della Commissione bilancio. Se questo è il contenuto, chiaramente anche io ed il collega Bordon non possiamo che essere favorevoli ad un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare quello che la Commissione bilancio sul punto ha deciso. Anticipo quindi il nostro voto favorevole.

di trasformare l'ordine del giorno che aveva un senso politico evidente in pura acqua fresca. Il Gruppo UDC non ha una posizione definita, perché di fronte all'acqua fresca è difficile decidere di votare a favore o contro. Ognuno dei colleghi vota come vuole.

l'articolo 8-*bis*, che viene sottoposto adesso alla valutazione definitiva dell'Aula, riproduce un emendamento che, come tutti sappiamo, è stato presentato

perché nell'approccio che la manovra finanziaria faceva complessivamente al problema dei costi della politica (con l'articolo 8, che abbiamo già votato e che scollega l'automatismo previsto per i parlamentari; con l'articolo 14 che incideva sulle rappresentanze locali, Consigli comunali e provinciali; con l'articolo 91, che intendeva calmierare i limiti di retribuzione previsti per la pubblica amministrazione), c'era chiaramente un vuoto: un vuoto: il Governo immaginava di intervenire trasversalmente su tutta la filiera per razionalizzare e contenere i costi della politica evitando un unico tasto, che era proprio quello del Governo. Ecco perché, fra le ragioni che abbiamo già espresso, ha sicuramente indotto diversi Gruppi a proporre questo emendamento quella di fare in modo che questo sacrificio, questo contenimento, questa razionalizzazione, sia esternamente sia internamente al Palazzo, fosse assolutamente coerente. In questa logica è stato presentato l'emendamento che si è poi tradotto nell'articolo 8-*bis* che viene ora posto al voto dell'Assemblea. Il ministro Mastella ha espresso delle perplessità,

al ministro Mastella - che non mi ascolta e continua a non ascoltarmi - vorrei ricordare che tutto il Governo ha preso atto che sostanzialmente questo emendamento reintroduce le norme previste dalla legge Bassanini

si accetta che si discuta della struttura del Governo. Noi non vogliamo discutere della struttura del Governo, abbiamo voluto reintrodurre una norma che conteneva, razionalizzava, norma che purtroppo, l'ho già detto...

...era stata abrogata una prima volta in occasione dello spacchettamento da parte del Governo di centro-destra nel 2001. Quindi, i primi che hanno violato quella norma, che conteneva delle regole precise rispetto all'amministrazione dello Stato,

non è giusto discutere della struttura del Governo perché noi ragioniamo di una corretta e razionale organizzazione del Governo, di un modello che abbiamo già discusso, deciso ed accettato nella passata legislatura. Lei poi, signor Ministro, ha affermato

che esiste una struttura di Governo esagerata. Allora, signor Ministro, se c'è questa consapevolezza anche da parte sua e se questa consapevolezza, per fortuna, è stata recuperata pure dal Governo, è evidente che una norma come l'articolo 8-*bis* ha diritto di cittadinanza, tecnicamente perché reintroduce una norma già esistente e politicamente perché ci auguriamo che il Governo, al di là della data di entrata in vigore della norma, prenda atto di una volontà che d'altra parte, se dichiara di condividere, deve dimostrare di accettare e condividere fino in fondo. Ecco perché, a nome mio e del collega Bordon, rappresento la volontà del voto favorevole all'articolo 8-*bis* che è stato sottoposto alla nostra valutazione.

Che si sia di fronte ad un attacco proditorio alle istituzioni mi sembra del tutto evidente; potevano pure rivolgersi a lei, piuttosto che al Presidente della Repubblica, perché è qui che si discuterà quell'emendamento.

Il mio partito è disponibile a rinunciare al proprio nome e al proprio simbolo subito. Chiediamo all'UDC di fare altrettanto e lo chiediamo anche a questi sedicenti proprietari del simbolo che vorrebbero utilizzarlo per rubare i voti all'UDC e a noi, visto che hanno un simbolo identico. È una vergogna! Mettiamo il simbolo nelle mani della fondazione don Sturzo cosicché nessuno lo potrà più utilizzare. Vedrà cosa le risponderanno questi sedicenti imbroglioni che vorrebbero prendere i voti dei cittadini ai danni nostri e dei democristiani.

infatti, dà il senso della nostra convinzione che una strategia incisiva debba oggi partire, per essere convincente e per essere capita dal Paese, dai rami alti. introduciamo regole più o meno stringenti per il contenimento e la riduzione dei costi della politica su vari livelli istituzionali. Sarebbe stato e sarebbe, a nostro avviso, un gravissimo errore limitarsi alle istituzioni minori, toccare i consigli circoscrizionali, le comunità montane, i consigli comunali, senza capire che è necessario dare un segnale forte anche per il più alto livello delle istituzioni.

Ricordo che già quando il Governo Berlusconi operò il primo spacchettamento, a tutti noto, fu aspra la polemica, così come è stata aspra quando il Governo Prodi ha proseguito sulla medesima strada.

E specificamente, per quanto ci riguarda, certamente non ha mai inteso essere, né intende esserlo oggi nel dichiarare il nostro voto favorevole, un'iniziativa contro il Governo in carica. Ho personalmente preso la parola in sede di discussione generale per spiegare i motivi di conformità a Costituzione che imponevano di non porre termini alla norma che ci accingiamo a votare, motivi che confermo con le medesime osservazioni che sono state ricordate anche nel dibattito di stamattina. Naturalmente, che il Governo debba poi valutare l'accaduto dal punto di vista politico è ovvio. Abbiamo approvato un ordine del giorno che richiede questo, ma anche se non lo avessimo approvato sarebbe stato ugualmente vero. È però che dal punto di vista sia formale che sostanziale si lasci alla dialettica politica la valutazione e la determinazione dei successivi esiti, nel confronto fra le parti politiche, nel confronto tra le sedi istituzionali

Lo dico soltanto perché la Costituzione e la buona politica lo impongono. Penso che l'iniziativa proposta in Commissione bilancio e da questa approvata sia stata avanzata, come è stato oggi ricordato, nella sede propria.

e addirittura - in alcuni casi, in certi articoli, in taluni emendamenti che sono stati approvati - in maniera retroattiva), quando si tratta di assumere una decisione di questo tipo, rinvia al prossimo Governo o comunque la rinvia. Di fronte a questo atteggiamento, il Gruppo di Alleanza Nazionale non potrà che votare contro l'articolo 8-*bis*.

auspicando (questo messaggio deve arrivare ai tanti amici che fanno parte della maggioranza) che siano rispettate anche le nostre idee

che non solo scarica i suoi effetti su un futuro Governo, ma scarica anche le coscienze di coloro che hanno sempre sostenuto la necessità di ridimensionare il Governo e che su questo punto hanno fatto la loro fama politica.

di giustificare da un punto di vista quasi costituzionale questa formula bizzarra, che rinvia al futuro Governo l'applicazione della norma, devono essere anche loro messi di fronte alle loro responsabilità. Infatti, non vi è stato alcun pudore costituzionale per i Governi insediatisi a decretare con urgenza la modifica della compagine ministeriale e a modellare poi base della nuova formulazione, mentre oggi vi sarebbe qualche *pruderie* di carattere costituzionale acché il Governo in carica rivedesse la propria compagine. Occorre anche coerenza coerenza e serietà e questo articolo non è coerente né serio per quanto è stato detto in questi mesi e in questi anni. Presidente, colleghi, voteremo contro questo articolo perché è assolutamente ipocrita. Ricordo che negli oratori che frequentavo da piccolo ironicamente sopra il banco del bar c'era scritto: «Oggi non si fa credito, domani sì». mi sembra che la logica di questo articolo vada nello stesso senso. In altri termini, il Governo che ha costruito l'Esecutivo più pletorico e numeroso della storia della Repubblica ritiene che un altro Governo, invece, dovrà essere snello. Contestualmente, l'Assemblea

alcuni dei quali - mi consenta di dirlo - sono dei fantasmi, perché nessuno li vede mai. Iniziate a dare il buon esempio voi: se aveste un minimo di coerenza, dovreste ridurre da subito il numero dei Ministri e dei Sottosegretari. Questo articolo aggiuntivo è dunque assolutamente inaccettabile. Signor Presidente, il Gruppo UDC voterà contro l'articolo per una semplice considerazione,

tra me e me, ma lo chiedo anche alla sinistra antagonista, quella che ha sfilato insieme ai precari e ai disoccupati:

che proponevamo con i nostri emendamenti, con i nostri ordini del giorno, dove vi invitavamo a prendere anche qualche mese di tempo ma a decidere oggi, perché il messaggio che mandate al Paese è che si possono, per fortuna poi non lo avete fatto, ma che si potevano ridurre i consigli comunali, i consigli provinciali, che si possono ridurre le comunità montane, che si possono bloccare le indennità parlamentari, che si possono bloccare tutti i costi della politica per gli altri meno che per questo Governo. Non è un messaggio positivo che si manda agli italiani, è un'ipocrisia. - mi consenta il collega Castelli - diventa una ipocrisia votare contemporaneamente un ordine del giorno che rimette la decisione alla competenza del Ministero del Ministero e poi votare contro l'articolo. Bisogna essere persone serie: noi dell'UDC vogliamo essere coerenti e persone serie e perciò votiamo contro l'articolo

anche la nostra componente voterà contro l'articolo 8‑*bis* per le motivazioni che sono state espresse più autorevolmente di me dai colleghi dell'opposizione. Aggiungo però un elemento. Lei che l'opposizione - stando almeno alle parole che ascoltiamo ogni giorno - si batte affinché questo Paese posso tornare alle elezioni e quindi avere un nuovo Governo. È un'opinione, la nostra, che che credo abbia diritto di cittadinanza. Dall'altra parte probabilmente si tenterà di ritardare questo momento e magari ci potrebbe essere la scappatoia di un nuovo Governo.

non si dovesse andare alle elezioni e ci dovesse essere un nuovo Governo, con tutti i passaggi istituzionali, la fiducia, vi avvisiamo, non ci si azzardi a fare votare requisiti di necessità e urgenza su un nuovo decreto che dovesse fare piazza pulita di questa norma. Lo dico perché il collega Villone da questo punto di vista è esperto: noi approviamo una norma, arriva un decreto che reistituisce i Ministeri, si stabilisce che c'è necessità e urgenza. Oggi la parte presuntamente maggioritaria del Parlamento - quella che è minoritaria nel Paese

signor Presidente, spero che ci sia grande vigilanza da parte della Presidenza del Senato, a meno che non diventi lei Presidente di quel Governo... PRESIDENTE. Grazie. La rivolga al Presidente del Senato la raccomandazione. Va bene

spero che abbia lo stesso diritto di cittadinanza delle opinioni espresse dai colleghi del centro-destra, che condivido. Abbiamo approvato a inizio legislatura e ricordo ancora che lei fece passare l'interpretazione - in questo caso lei - sulla nostra richiesta di votare per parti separate i presupposti di costituzionalità sul decreto riguardante lo spacchettamento dei Ministeri, ci fece dividere i Ministeri sull'onda della volontà del Governo. Il ministro di Pietro ci dice, un giorno sì e l'altro pure, che è uno scandalo che infrastrutture e trasporti siano divisi,

Come si suol dire, «carta canta e villan dorme», oggi con un voto a maggioranza si impegna in realtà la maggioranza di domani. Ci potrebbe essere la scappatoia di un nuovo Governo. Non ci si azzardi a cambiare questa norma per favorire ancora una volta la sinistra.

A nostro avviso, è opportuno indicare un altro punto, ovvero quello delle liquidazioni, non solo quelle scandalose di centinaia di milioni di euro, ma anche quelle di rappresentanti del pubblico in enti e in società

se il senatore Rossi accettasse la votazione per parti separate, noi potremmo votare a favore della seconda parte dell'ordine del giorno in titolo. Approfitto di avere la parola perché purtroppo io sono un leghista e non sono aduso ad accettare le provocazioni,

con l'augurio che possa essere condiviso e votato da questa Assemblea. Nel periodo estivo abbiamo assistito a molte iniziative, alcune delle quali purtroppo più propagandistiche che operative, come quella del sindaco di Firenze sui lavavetri, che hanno segnalato come ci sia l'esigenza anche da parte degli enti locali di poter aumentare il proprio intervento rispetto alla sicurezza reale e percepita da parte dei cittadini.

come la videosorveglianza, o in quanto altro possa essere utile ad aumentare la sicurezza dei cittadini. Escludere le maggiori spese, sia per parte corrente sia per parte investimenti, dal Patto di stabilità interno sarebbe di grande aiuto alle amministrazioni locali per assumere iniziative concrete a vantaggio della sicurezza dei cittadini. Se i colleghi di ogni parte politica davvero credono a quello che spesso dicono, ossia l'interesse dei cittadini ad avere maggiori interventi verso la sicurezza, non possono che prendere in considerazione la possibilità di votare in modo favorevole a questo emendamento.

locali, magari sindaci, assessori o consiglieri comunali, di sostenere questo emendamento per poter affrontare più efficacemente il problema della criminalità, come ha giustamente detto poc'anzi il collega Fluttero.

Anche il Governo esprime contrarietà, ma, molto sinteticamente, vorrei ricordare che il Patto di stabilità, essendo fondato il Patto di stabilità, essendo fondato sui saldi di bilancio, lascia intatta la sovranità del singolo ente in merito alle priorità che vuole perseguire con la propria politica di spesa. Pertanto, da questo punto di vista non c'è alcun vincolo, se non il rispetto del vincolo di bilancio complessivo.

di illustrare questo emendamento, ma perché l'argomento è particolarmente complesso, a volte di difficile comprensione, e richiede quindi da parte nostra un piccolo sforzo, nella corsa che stiamo facendo in questi giorni per approvare la legge finanziaria, che ci consenta di approfondire per alcuni minuti un tema che si sta dimostrando ben più difficile di quanto potessimo immaginare. Non tutti i colleghi senatori hanno esperienze o competenze di finanza e, quindi, spero di poter essere molto chiara e di riuscire a trasferire a ciascuno di noi alcuni semplici concetti che ci aiutano a meglio comprendere cosa sta accadendo nel nostro Paese, in relazione a processi finanziari sempre più difficili da comprendere, non solo per la complessità della materia, ma anche perché,

poco trasparenti - anzi, vorrei dire così opachi - da rendere difficile a chiunque, anche a grandi esperti di finanza, la capacità di valutare alcune mirabolanti operazioni che nel nostro Paese stanno determinando

ad un convegno, ha espresso forti preoccupazioni sul tema dei derivati - perché è di questo che parliamo - che da qualche tempo rende nervosi clienti ed investitori delle banche italiane. Greco risulta che in Italia i derivati stipulati dalle pubbliche amministrazioni ammontino a ben 13 miliardi di euro e questo gli fa dire che ci troviamo in un mondo in cui ricchezza e perdite sono fuori da ogni trasparenza e, quindi, da ogni controllo e che questa situazione potrebbe riflettersi su di noi con una possibile crisi.

ahimè, nessuna competenza consente di comprendere realmente quali sono i costi veri che la banca chiede di pagare nel momento in cui l'ente locale sottoscrive il contratto. I costi impliciti,

per poter individuare chi si assume la responsabilità, e in qualche caso la colpa grave, di aver nascosto all'ente locale alcune valutazioni riferite ai costi, ma non solo, che invece dovevano essere chiaramente individuate. nel corso dell'*iter* di questa finanziaria tanti di noi, della maggioranza e dell'opposizione, hanno condiviso la forte necessità di di riscrivere le regole di questi derivati. Per fare ciò nel migliore dei modi abbiamo la necessità però di conoscere questo fenomeno. Apprezzo molto l'iniziativa di Bankitalia che ha avviato delle indagini in tal senso, facendo comprendere a tutti noi che quel rischio c'è, eccome, e che

da legislatori al Paese intero strumenti di maggiore trasparenza, ma anche di maggiore rispetto delle regole. Vede, signor Presidente, gli enti locali ormai, a forza a forza di fare simili operazioni, hanno accumulato un debito fuori da ogni controllo. Questo ci deve preoccupare, ci deve preoccupare, e molto. Per arrivare ad una conclusione più rapida anche in questa finanziaria, la nostra proposta è quella di non fermarsi all'emendamento che il Governo ha proposto, ma di fare uno sforzo in più per aggiungere a quell'emendamento alcune forme di garanzia e di tutela che consentano a tutti noi di stipulare serenamente con le banche italiane,

dopo un pronunciamento della Camera dei *Lord*,in Inghilterra quei prodotti non possono essere proposti agli enti locali? Perché si consente che il nostro Paese sia terreno di *shopping* selvaggio da parte di banche straniere che rischiano di mettere in crisi le banche italiane, ma soprattutto il nostro sistema degli enti locali che tra un po' sarà completamente ostaggio degli enti locali stessi? Per questo chiedo un voto

sta suscitando una grande attenzione nell'opinione pubblica, abbiamo svolto una discussione approfondita in Commissione e abbiamo approvato il testo

luogo che i contratti cosiddetti derivati siano informati alla trasparenza. Questo testo è identico al testo Bonfrisco. Secondo, che i contratti derivati rechino le informazioni che saranno fissate con un decreto del Ministro dell'economia, sentiti CONSOB e Banca d'Italia. Anche sotto questo profilo, il testo è analogo a quello della senatrice Bonfrisco. Dopodiché stabiliamo che il Ministero dell'economia dovrà verificare la corrispondenza tra i contratti che saranno stipulati dagli enti locali e dalle Regioni ed i modelli in tal modo predisposti ed approvati e dopodiché stabiliamo che il rispetto di queste condizioni costituisce elemento costitutivo dell'efficacia del contratto. Se non si rispettano queste regole il contratto è nullo.

superato il quale, il rischio stesso ricade sugli operatori finanziari, sulle banche che propongono quei prodotti e su pochi altri. condivido l'esigenza di ripartire il rischio, purtuttavia da chi è più esperto di me e di noi ci viene fatto rilevare che questa costituirebbe una seria e invasiva violazione dell'autonomia negoziale delle parti contrattuali; si andrebbe ad incidere sulla volontà contrattuale, che, ripeto, con il testo approvato viene comunque incanalata dentro binari che saranno ben definiti con il decreto che emanerà il Ministero dell'economia. Per queste ragioni esprimo parere contrario,

Signor Presidente, data la rilevanza dei temi, al di là del conformarmi al parere del relatore, vorrei comunque svolgere un breve commento. Innanzi tutto vorrei ricordare come su questa delicata ed importante tematica è stata proprio l'iniziativa del Governo dello scorso anno, che è stata poi approvata dal Parlamento, ad avviare questa serie di attività che hanno consentito anche di far emergere alcune situazioni critiche. Vi è piena condivisibilità sulle finalità che si vogliono raggiungere con l'emendamento 10-*bis*.800. Vi sono invece alcune perplessità in merito gli strumenti che si vogliono utilizzare per raggiungere tali finalità. Vorrei ricordare come, per esempio a proposito dei prospetti informativi, vi siano delle direttive comunitarie che individuano con precisione i temi che debbono essere affrontati dai prospetti in merito all'eventuale

ma non dell'introduzione di vincoli contrattuali, che, come ha ben ricordato anche il relatore, lederebbero l'autonomia contrattuale delle parti. Per tale ragione, come

su questa vicenda, perché non è così innocente e natalizia la distanza tra la posizione del Governo e quella espressa dai firmatari di questo emendamento. intanto al sottosegretario Sartor che nella direttiva europea che riguarda le tipicità di trasparenza che debbono apparire nei contratti non c'è nulla che contraddica ciò che propone in questo momento la collega Bonfrisco.

per mettere in sicurezza gli enti locali di fronte ai problemi che possono scaturire da un'errata gestione degli strumenti riconducibili

sottoscrittore dello strumento finanziario devono attestare espressamente di aver preso in considerazione. Quindi, è prevista un'autocertificazione della consapevolezza di ciò che si è fatto in questa norma, che francamente muove poco la classifica dal punto di vista delle sicurezze da acquisire su questo tipo di operazioni.

benefico per gli enti locali e per le Regioni - ci sono state delle cadute che hanno mostrato il rischio di questo tipo di operazioni e l'inconsapevolezza con cui in esse ci si avventura, spesso e volentieri, su istigazione di *broker* molto spregiudicati. Approvare questa norma significa arrivare alla Camera con una situazione più chiara sul livello dell'intervento che il Parlamento intende attuare su simili questioni, non votarla significa affidarsi, mani e piedi legati, a quello che deciderà il Governo. Alleanza Nazionale sceglie di cominciare a decidere da adesso. EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, non è esatto quello che ha detto il Sottosegretario: è l'opposizione che, con la sua azione, ha determinato le condizioni per far emergere il quadro complessivo dei derivati e lo ha fatto in Commissione. Chiedo, anzi, alla senatrice Bonfrisco di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento. Abbiamo posto il problema della trasparenza. Il testo della Commissione è un passo avanti, ma insufficiente, perché gli enti locali si sono avventurati sul terreno della scommessa, si sono fidati di intermediari finanziari, ma chi vende sa che cosa vende, compra, e gli enti locali non lo sapevano. C'è una parte di enti locali che ha fatto operazioni addirittura sui mercati internazionali, che sfuggono anche al controllo della Banca d'Italia e quindi non emerge un quadro complessivo di questo fenomeno. Riteniamo

che la sottostima da parte del Governo di questo fenomeno è assai evidente, e ha ragione il senatore Eufemi: il relatore Legnini ha il grande merito di aver tentato di trovare una formula che consentisse non solo alla Commissione bilancio, ma all'intero Senato una soluzione per cui i rappresentanti dei cittadini chiedano al Governo e impegnino il Governo, attraverso un dispositivo di legge, a fare quello che il Governo finora non ha fatto. So bene, che non è solo il Governo che avrebbe dovuto fare qualcosa. Mi piacerebbe sdrammatizzare l'aria attorno a questo fenomeno che invece è assai triste: c'era una nostra collega, qualche tempo fa, che alla domanda:

quale vigilanza abbia operato la CONSOB su questo fronte. Ahimè, ritengo sia quella stessa che ha operato quando ha affrontato i casi Parmalat e Cirio,

che abbiamo sottoscritto in tanti di noi della Casa delle Libertà, ma di aprire gli occhi e di garantire quei cittadini che, invece, in questo Governo non trovano nessuna garanzia. molte banche trovano molte garanzie in questo Governo, ahimè, quasi tutte straniere. Questo è il vero tema sul quale dobbiamo ragionare: se questo Governo è in grado di garantire la sicurezza non solo fisica ma anche dei risparmi dei suoi cittadini, oppure no.

la questione non è stata esperita. Se la questione sta nei termini posti dal relatore, e cioè che tanti punti sono in comune, tralasciando le considerazioni politiche della senatrice Bonfrisco che vanno al di là del contenuto dell'emendamento, il timore del relatore è che si vada ad invadere una competenza delle banche. Credo che il Senato ne abbia tutte le facoltà dovrebbero essere le banche a non invadere, come stanno facendo, la vita economica e politica di tutti gli italiani. Quindi, io voterò a favore dell'emendamento

Signor Presidente, condivido l'impostazione data dalla senatrice Bonfrisco, con cui abbiamo anche Prendo anche atto, però, delle dichiarazioni sia del relatore che del Governo in relazione alla politica che si intende fare per garantire i risparmiatori e i nostri enti locali. Annuncio, quindi, il mio voto di astensione

Va bene. È evidente che c'è un parere diverso tra la senatrice Bonfrisco e il presidente Morando. Non avendo altre richieste di intervento, pregherei i colleghi di prendere posto, perché dobbiamo procedere al voto. Ci saranno alcune votazioni

la dichiarazione di voto

una grande e forte voglia da parte di questo legislatore di intervenire (a piè pari, sistematicamente e in maniera molta pesante) su argomenti che invece attengono alle amministrazioni locali, le quali assolutamente non possono essere accomunate ai ai risparmiatori - poveretti! - che devono essere assolutamente tutelati. Gli amministratori locali sono eletti dal popolo a suffragio universale e dovrebbero essere competenti; dovrebbero intervenire nel predisporre strumenti finanziari che fanno parte dell'economia moderna, che sorreggono, al pari delle attività produttive, tutto il mondo economico. È come se oggi dovessimo rinunciare ad utilizzare Internet, perché è uno strumento moderno che non si capisce. Non è così. Lo strumento finanziario dei derivati sostiene l'economia moderna al pari delle attività produttive. Se ci sono delle deformazioni e delle distorsioni, gli gli amministratori locali dovrebbero avere la competenza e il buon senso di saper amministrare i propri enti locali e quindi di predisporre adeguatamente Lo fanno attraverso dei semplici strumenti di conoscenza. Vorrei solo rammentare che spesso il presidente della Provincia, piuttosto che il sindaco, utilizza il derivato consapevole del fatto che abbassando la rata nell'immediato futuro salverà la propria legislatura e rimanderà ad un futuro più lontano la necessità di rientrare di quel debito. Ma questo non può essere regolato per legge; questa valutazione

della pubblica amministrazione e dell'amministrazione locale dovessimo fare quello che stiamo per fare nel campo della finanza, dovremmo regolare dettagliatamente ogni azione dell'ente locale.

l'interesse e l'impegno che alcuni colleghi hanno messo nel corso del dibattito sulla finanziaria attorno a questo problematica. In particolare, do atto alla senatrice Bonfrisco di essersi impegnata al massimo per richiamare l'attenzione su una problematica seria, complessa e difficile. però qualcuno ha detto, occorre fare attenzione ai confini che dobbiamo porci attorno ad una polemica che certamente ha il diritto di essere svolta. Occorre sapere che il sistema dei derivati oggi è parte strutturale del sistema finanziario italiano, europeo e mondiale. Sarei più dell'avviso che queste problematiche

riguarda il sistema creditizio e finanziario è uno dei più avanzati d'Europa e coloro che contestano simile affermazione evidentemente non sono né documentati, né aggiornati. Quindi, se si vuole affrontare in maniera organica, puntuale, ancora più precisa, mettere dei paletti, ulteriori controlli, attorno a queste emissioni, per carità, lo si faccia, ma senza per questo buttare l'acqua sporca con il bambino dalla finestra. Quindi, anch'io, signor Presidente, mi asterrò

13. I nostri lavori proseguiranno sulla legge finanziaria sino alle ore 13. A questo punto, però, la Presidenza decide di anticipare la ripresa dei lavori questo pomeriggio dalle ore 16 alle ore 15,30, restando fissato il termine della conclusione 19. Pregherei i colleghi, anche in relazione a questo ulteriore accorciamento dei tempi, di accelerare molto nei loro interventi i giudizi e le valutazioni su emendamenti e su articoli di legge, perché siamo gravemente in ritardo rispetto alla tabella di marcia che era stata prevista e prefissata.

Signor Presidente, voterò contro questo articolo, non perché sia affezionato al tema dei derivati, ma perché sono affezionato alla Costituzione e all'autonomia degli enti locali. Questo articolo - così come molti altri, sui quali avrò la possibilità di intervenire brevemente nel prosieguo del dibattito - rappresenta un pericoloso quanto incostituzionale attentato all'autonomia e alla responsabilità degli enti locali. Il vero pericolo dell'attività finanziaria impropria che alcuni enti locali hanno messo in piedi, signor Presidente, colleghi, è il successivo intervento del Governo, così come è avvenuto con il precedente decreto fiscale, quando si sono impiegati 150 milioni di euro per risanare i bilanci di Comuni che avevano male amministrato. Allora, se è vero che bisogna dare moralità al sistema al sistema finanziario degli enti locali, lo si deve fare con gli strumenti appropriati e non con questo tipo di interferenza impropria nella loro autonomia. Rispettiamo il Titolo V della Costituzione, se lo conosciamo,

la possibilità di utilizzare le spese di progettazione regolando i rapporti con il proprio tecnico e potendo iscrivere nelle loro partite tali tali entrate per il funzionamento dell'ente locale. Quindi, un piccolo Comune, invece di andare a progettazione esterna, iscrive nel progetto europeo le spese di progettazione e le introita,

cominciare a seguire un'altra via e non lasciare che le cose vadano avanti come sono andate avanti finora. L'anno scorso avevamo previsto alcune misure in finanziaria che mi pare tuttavia

Presidente, il Gruppo dell'Ulivo, conformemente a quanto espresso dal relatore e conformemente al parere del Governo, esprime un voto contrario a questo emendamento. Certo, il blocco delle assunzioni nei grandi Comuni, con la definizione di un rapporto tra dipendenti e residenti, crea oggettivamente dei problemi che

*(LNP)*. Signor Presidente, ormai siamo insieme da un anno e mezzo e abbiamo fatto migliaia di votazioni. Sono molte centinaia di volte che il senatore Garraffa ci tormenta, o quanto meno tormenta

costi». Con l'emendamento 13.1 proponiamo di sopprimere questo articolo perché riteniamo che l'articolato, così come è stato definito dai passaggi in Commissione, non risponda agli obiettivi di razionalizzazione, né di contenimento dei costi. Riteniamo sia decisamente più opportuno che questo articolo rimanga inserito a pieno titolo nella discussione del codice delle autonomie locali (discussione, peraltro, aperta da mesi),

Questi sono alcuni dei motivi, emersi da un'attenta lettura del testo così come viene proposto all'Aula, che confermano quanto si sosteneva all'inizio, cioè che questo provvedimento non razionalizza, anzi rischia di creare ulteriore confusione in un settore abbastanza complesso. C'è poi l'aspetto del "contenimento dei costi" che viene citato nella rubrica di questo articolo. Ben venga il contenimento dei costi, ma solo se è reale,

e questi risparmi sovradimensionati non vengono utilizzati per obiettivi virtuosi. Basta scorrere rapidamente l'elenco delle spese discutibili che sono inserite in finanziaria. Ve ne leggo alcune: 2 milioni di euro di fondi per l'apicoltura all'articolo 29-ter; 50 milioni di euro per aree verdi in zone urbane all'articolo 45 (potrebbero tranquillamente

personale del pubblico impiego è contrario all'obiettivo di riduzione dei costi nella pubblica amministrazione. Concludo la mia breve digressione sul personale della pubblica amministrazione,

di una formulazione dell'articolo 13 che non risolve il problema delle comunità montane, ma potremmo dire, con un gioco di parole, che in questo caso la montagna ha partorito il topolino. Tuttavia, il problema esiste e ci

il cosiddetto codice delle autonomie, i cui tempi di discussione e di esame da parte di questo ramo del Parlamento sono certamente destinati a prolungarsi notevolmente.

quando furono istituite le comunità montane, nel 1971, erano tempi di ristrettissime deleghe alle Province ed era anche una fase storica il cui il problema dell'abolizione delle Province del giorno. Negli anni successivi si è attuata una modifica nell'equilibrio delle competenze dei poteri locali: alle Province sono stati affidati compiti in materia di difesa del suolo, deforestazione, parchi, riserve naturali con funzioni che riassorbono quelle assegnate alle comunità montane. La sopravvivenza delle comunità montane, quindi, se non abbiamo il coraggio di affrontare il tema della revisione costituzionale e dell'abolizione delle Provincia, non ha più significato. È un costo aggiuntivo e una complicazione del nostro sistema di autonomie locali. Vorrei portare all'attenzione dei colleghi a sostegno della mia richiesta di sopprimere gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico degli enti locali. Oggi siamo in presenza di 356 comunità montane, la cui superficie è di 16 milioni di ettari, a fronte di superfici montane del Paese di soli 10 milioni di ettari.

Ma 111 milioni e 615 euro, indicati come spese in conto capitale, sono destinati all'amministrazione generale, alla gestione e al controllo. Se poi guardiamo alle tabelle relative alle spese per investimenti divise per interventi si accerta che per l'acquisizione di beni immobili sono stati spesi 353 e 665.000 euro su un totale di 862 milioni e 246.000 euro. Quindi, non siamo in presenza di spese di investimento ma di rilevanti spese per acquisizione di immobili o spese correnti. Se pensiamo che hanno 7.500 dipendenti, il 15 per cento di quelli delle Province, e che le spese per gli emolumenti dei presidenti delle comunità montane ammontano 13 milioni e 680.000 euro, mentre non abbiamo i dati per i gettoni dei consiglieri, ci rendiamo conto come questo rappresenti un costo della politica reale che non risponde più a funzioni

delle comunità montane sostituendo all'articolo 13 del testo del Governo la proposta di abolizione degli articoli 27, 28 e 29 del testo unico degli enti locali mi sembra meritevole del consenso dell'Aula.

che ci troviamo di fronte ad un problema troppo grande perché sia risolto nell'*omnibus* di una finanziaria. La riforma delle comunità montane va stralciata

come quello delle comunità montane potrebbe trovare un maggiore approfondimento, un'analisi seria ed una considerazione sulle ripercussioni che avrebbe. Signor Presidente, non voglio offendere nessuno. Non si possono giudicare le comunità montane vivendo in città. Bisogna capire cosa esse rappresentano ancora in determinate situazioni e località di montagna. È vero che vanno ridimensionate, modernizzate e ridotte, ma non si possono cancellare cancellare con un colpo di spugna incosciente come questo. Una delle conseguenze collaterali, non secondaria secondo me, è proprio quella che ha ricordato prima il collega Del Pennino, seppure con una intenzione opposta rispetto alla mia:

spendere qualche parola di motivazione. Su questo articolo, licenziato dalla Commissione bilancio e sostituivo di quello proposto dal Governo,

a regime; non incide né sull'autonomia degli enti, né sulla potestà legislativa delle Regioni che viene espressamente salvaguardata con l'indicazione di criteri, ai quali le Regioni devono attenersi nel ridisciplinare questa materia entro il 30 giugno. Voglio solo dire all'Assemblea che con questo articolo riduciamo

sottolineate anche dalla stampa e dall'opinione pubblica, ma non usando l'accetta nella ridefinizione dei territori di montagna perché sappiamo i problemi che si erano posti a seguito dell'indicazione rigida di quel criterio di ridefinizione della montanità proposto ma confermato come criterio dato alle Regioni, più attenuato ma nel contesto di un'operazione di razionalizzazione e di riduzione, risparmio vero sui costi della politica. Infine, relativamente a questi risparmi abbiamo migliorato sensibilmente il Fondo per la montagna, confermando i 50 milioni proposti dal Governo nel testo originario e aumentando quello previsto nel secondo e terzo anno da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro. Faccio notare all'Assemblea che il Fondo della montagna, fino all'anno scorso, era stato fissato in 25 milioni di euro e che nel passato Governo era stato totalmente o

il parere del Governo in merito agli emendamenti è conforme a quello del relatore. Circa l'ordine del giorno G13.100 il parere è favorevole come raccomandazione,

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire anzitutto per evitare ai colleghi una confusione, perché il relatore, nel dare il parere, è arrivato

sottoscrittori dell'emendamento soppressivo 13.1 di ritirarlo, per poi confluire sulla votazione contraria dell'articolo 13. Mi sembra infatti di ricordare, a termini di Regolamento, che l'eventuale bocciatura dell'emendamento soppressivo precluderebbe gli altri emendamenti e soprattutto la votazione sull'articolo, che è quella fondamentale. Quindi, se i sottoscrittori

se poi lo sbocco sarà quello che ha detto il collega D'Alì, che porterà ad un voto contrario

colleghi, sia della maggioranza che dell'opposizione, avevamo presentato un subemendamento all'emendamento del relatore in Commissione bilancio che per me ancora costituisce un punto di riferimento valido.

di aver fatto un passo in avanti rispetto al testo del Governo, perché le risorse vengono mantenute alla montagna. C'è però un problema sul quale secondo me la Camera dovrebbe essere invitata a ritornare, anche per cercare di comporre meglio il rapporto con la montagna.

dovrà prevedere per tutto il territorio nazionale come unioni, per me obbligatorie, di Comuni sotto una certa dimensione demografica. Non si può pensare di abrogare un centinaio di comunità montane ponendo i costi dei servizi da queste resi a carico dei Comuni che ne fanno parte. Bisogna mettere mano alla classificazione dei Comuni montani, a cui il senatore ha anche fatto riferimento, con la nuova legge sulla montagna o con la modifica della legge sui piccoli Comuni; in questo senso, è giusto ridurre, come ha detto il relatore, senatore Legnini,

abbiamo cercato di essere assolutamente coerenti con la sostanza degli argomenti più che con l'apparenza. Voterò a favore della soppressione di questo articolo, perché mi meraviglia che il Governo, il relatore e tanti illustri colleghi che hanno esperienza di diritto costituzionale possano pensare che questo emendamento non intervenga a stravolgere i principi essenziali del Titolo V della Costituzione e dell'ordinamento degli enti locali. Tra l'altro, il codice delle autonomie è all'attenzione delle Commissioni parlamentari perché è lo stesso Governo che lo ha proposto. Come si fa adesso in finanziaria ad intervenire dicendo delle assurdità? La prima cosa corretta che si dice - l'unica - è che le comunità montane sono da intendersi (ma anche questa è una novella legislativa) come Unioni di Comuni. Tutti noi sappiamo che le Unioni di Comuni sono momenti di aggregazione volontaria dei Comuni. Quindi, il fatto che si dica che le comunità montane sono Unioni di Comuni mi sta bene, perché rispetta certamente l'autonomia degli enti locali nella decisione di aggregarsi tra loro per dare servizi in collettività ai cittadini. viene subito dopo smentito nel momento in cui l'articolo riconferma la prassi attualmente in essere - a mio giudizio assolutamente incostituzionale - che siano le Regioni ad individuare le comunità montane. Delle due l'una: o le Unioni di Comuni nascono come spontanee aggregazioni di Comuni, o sono le Regioni che decidono sulle comunità montane. Si arriva però all'assurdità di confermare per le Regioni la possibilità di obbligare

in un paradosso di incostituzionalità e mi meraviglia che colleghi così avveduti - come ormai da tanti anni ho avuto modo di apprezzare in questo Parlamento, che fanno parte della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali - non abbiano

nell'ambito del territorio comunale e che questo faccia scattare la qualifica di Comune montano (e ciò potrebbe al limite essere compatibile con una norma d'intervento statale) ma addirittura che questo Comune montano possa fare o meno parte di una comunità montana che viene qualificata come Unione di Comuni (cioè come aggregazione spontanea di Comuni), ma che poi questo sia stabilito con decreto del Presidente della Regione.

una maggioranza consimile a quella che oggi governa il Paese che però smentisce sé stessa dal momento che, dopo aver affermato una buona legge di principio sull'autonomia degli enti locali, la va a smentire clamorosamente stabilendo un centralismo peggiore di quello stabilito da Ricasoli nel 1861.

Presidente, vorrei sapere se il senatore Del Pennino, che è del mio stesso Gruppo, rappresenta la dichiarazione di voto del Gruppo,

Devo ammettere che qualche cosa è stata migliorata dagli emendamenti successivi. Non è ancora quello che chiedevamo. Quindi, il dispositivo può servire in effetti per colmare alcune lacune. Per esempio, è giusto il no ai Comuni costieri e ai capoluoghi di provincia, ma rimane come elemento su cui non siamo ancora d'accordo l'indice unico di valutazione della montanità riferito all'altitudine, come rimangono ancora molte perplessità

ordinamentale in un documento di bilancio, e sembra che questo - me lo insegnano i professori presenti - non sia possibile. Inoltre, non è ancora soddisfacente la disponibilità per il Fondo nazionale della montagna. Tuttavia,

inoltre gradito che il parere del Governo fosse stato espresso dal Ministro per gli affari regionali, che ha presentato il nuovo codice delle autonomie che va ad incidere su questa materia, la quale, purtroppo, non ha potuto partecipare alla discussione

che vengono eliminate per i consiglieri comunali, mentre un'altra parte riguarda la moralizzazione nella corresponsione dei gettoni di presenza, nel senso che i regolamenti comunali devono stabilire norme che certifichino e verifichino l'effettiva presenza alle riunioni. L'ultima norma riguarda

Presidente, anche per questo articolo la Commissione ha svolto un lavoro molto approfondito, pervenendo ad approvare una norma, un articolato interamente sostitutivo di quello in origine proposto dal Governo, e cioè stralciando la norma di riduzione del numero dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali (tema che si è ritenuto di dover demandare alla riforma *in itinere* del codice codice delle autonomie). In sostanza, si sostituisce questo articolato con una serie di norme che non incidono, come è stato erroneamente detto, sull'unità di misura del gettone di presenza dei consiglieri comunali, provinciali o degli assessori o dei sindaci. Infatti non tocchiamo l'entità dei gettoni di presenza delle indennità, ma vogliamo incidere, in misura anche significativa, sui meccanismi che a volte determinano anomalie nel

che, per esempio, fanno divieto di forfetizzare il gettone di presenza in una indennità mensile, da parte dei consiglieri comunali, provinciali, e così via. È vero che si riduce il tetto del compenso massimo da un terzo al 25 per cento di quello del sindaco, ma è altresì vero

non sia più riferita ai commi 18, 19, 20, 22 e 23, ma ai commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. La sostanza è identica ma la proposta è meglio formulata sotto il profilo tecnico. Rinnovo naturalmente in questa occasione la richiesta al relatore e al Governo

Come precedentemente comunicato, dopo l'intervento del rappresentante del Governo ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti ed il Gruppo Misto dieci minuti. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, dottor Naccarato. NACCARATO, *sottosegretario di Stato Signor Presidente, onorevoli senatori, sono qui a riferire sul tragico incidente che ha causato il decesso di sei militari americani ed il ferimento di altri cinque loro commilitoni, tutti in forza alla Compagnia G del 52° *aviation regiment* dell'esercito degli Stati Uniti di stanza ad Aviano. In questa dolorosa e triste circostanza, desidero innanzitutto esprimere, a nome del Governo e delle Forze armate italiane, le più sincere e profonde espressioni di partecipazione e cordoglio ai familiari delle vittime ed alle Forze armate statunitensi per il grave lutto che li ha colpiti. Passo subito all'esposizione dei fatti così come sono stati ricostruiti sulla base delle informazioni sinora pervenute. ore 12,25 circa di ieri mattina, un elicottero da trasporto tattico UH60 *black hawk*, con a bordo 11 militari decollato alle ore 11, 40 locali dalla base militare di Aviano, sede del 52° *aviation regiment* dell'esercito americano, mentre effettuava un volo di addestramento regolarmente pianificato, che prevedeva il sorvolo dell'area del fiume Piave ed il rientro dopo due ore circa, precipitava al suolo durante una manovra sulla zona di Grave del Piave, nel comune di Spresiano. Nell'impatto perivano quattro militari, mentre gli altri sette occupanti riportavano ferite varie; di questi, tre versavano in gravissime condizioni. Successivamente, in ospedale, nelle ore seguenti decedevano ulteriori due militari. Al momento dell'impatto le condizioni meteorologiche erano buone e non è stato segnalato il coinvolgimento di terzi né danni a cose. L'elicottero non trasportava alcun tipo di armamento e di munizionamento. Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i soccorsi (carabinieri, anche con elicotteri del 14° nucleo di Treviso, Eliambulanza, volontari del soccorso alpino, Vigili del fuoco e Polizia di Stato) ed i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Treviso, Castelfranco Veneto e Padova. La magistratura, ordinaria e militare, è stata informata così come le autorità americane.

Signor Presidente, l'incidente dell'elicottero militare che si è consumato ieri lungo il greto del fiume Piave nella zona di Santa Lucia, vicino a Conegliano, in provincia di Treviso, ha avuto purtroppo, come ci ha appena confermato il Governo, un bilancio tragico che sarebbe potuto essere ancora più grave data la vicinanza del punto dell'impatto ad un tratto autostradale. Esprimo, anzitutto, profondo cordoglio per le numerose vittime americane. Per quanto attiene, poi, alla dinamica, ci risulta che l'elicottero militare statunitense UH60 *Black hawk* stava eseguendo un volo di addestramento dopo essere partito dalla base militare di Aviano. Il programma di volo prevedeva un giro sulla zona e poi il rientro alla base nel pomeriggio. Dopo un'ora circa di addestramento, il velivolo si è avvitato su se stesso ed è precipitato. Ci auguriamo che le cause dell'incidente vengano presto chiarite dalla magistratura italiana, a mio avviso competente per territorio, e che il Governo possa acquisire ancora maggiori informazioni rispetto a quelle appena illustrate dal Sottosegretario.

che questi soldati sono presenti sul nostro territorio perché in un sistema integrato di difesa di un'alleanza internazionale essi garantiscono la libertà

che, invece, questa sia un'occasione per fare cattiva propaganda contro le nostre relazioni internazionali e contro il nostro sistema di alleanze. Ho già letto sui giornali che una serie di gruppi politici e di organizzazioni antagoniste alle alleanze militari storiche del nostro Paese

mesi, questo tipo di incidenti sarà destinato ad aumentare. Quello della sicurezza è uno degli elementi che si oppongono ad una progressiva militarizzazione del territorio e ad un affollamento di basi

la collega Valpiana. Non solo, in queste basi, per esempio ad Aviano, da cui è partito l'elicottero, e a Ghedi, abbiamo ordigni atomici, contro contro i trattati di non proliferazione che prevedono che solo gli Stati membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU possono possedere armi atomiche e questi stessi Paesi non possono cederle ad altri.

grave situazione, quella che avrebbe potuto provocare un incidente di questo genere su strade trafficate o su centri abitati, del resto ad abbastanza vicini. Non abbiamo elementi per fare fare valutazioni di altro tipo, nel senso che l'inchiesta USA-Italia non ha ancora prodotto alcun risultato, non ci sono elementi. Infine

onorevole rappresentante del Governo, mi unisco naturalmente al dolore e al cordoglio in vicinanza ai familiari delle vittime coinvolte nel tragico incidente di ieri; manifesto anche al Comando statunitense la sincera solidarietà e partecipazione mia personale e del Gruppo Per le Autonomie, nonché i più sinceri auguri di pronta guarigione ai feriti. Accanto a questo, tuttavia, c'è in noi una grande preoccupazione per le implicazioni dell'incidente, per quello che poteva essere e che, per fortuna, non è stato. Chiediamo che il Governo si faccia parte diligente per procedere a un'attenta verifica delle misure di salvaguardia e di prevenzione dei rischi per la nostra popolazione civile. Non si tratta di una questione ideologica, ma quella parte del Paese, quel territorio che conosco bene perché da lì provengo, è una grande città diffusa,

di pochi mesi fa anche lo schianto dell'aereo militare F16 a Zoldo Alto e questo incidente ci ha riportato anche alla memoria le scene della strage del Cermis. Cermis. Al di là di arroccamenti ideologici, vorrei veramente invitare il Governo, assieme alle autorità militari alleate, a riconsiderare l'opportunità di predisporre esercitazioni militari in zone così densamente abitate. Infine, c'è un aspetto giurisdizionale che vorrei evidenziare: benché il fascicolo aperto dal pubblico ministero trevigiano, Giovanni Cicero, sia per disastro aviatorio, l'azione penale spetterà alle autorità statunitensi, com'è successo due mesi fa per lo schianto dell'F16 a Zoldo Alto.

di Treviso rimane l'attività urgente, l'accertamento della dinamica, la conservazione delle fonti di prova e la nomina di un consulente, al quale si affiancherà quello di fiducia degli americani. Su questo aspetto mi sento di condividere quanto dichiarato dal parlamentare di Forza Italia, il collega Maurizio Paniz,

Mi auguro e sono fiduciosa che il Governo si farà carico di queste nostre richieste. Signor Presidente, a nome del Gruppo dell'UDC, esprimo anch'io un convinto cordoglio alle famiglie dei caduti, all'esercito americano e a tutta la nazione americana. Porgo un augurio ai feriti per una pronta guarigione. Si è trattato - lo ha ricordato bene il rappresentante del Governo - di un incidente che può rientrare nel novero delle probabilità all'interno di esercitazioni che avvengono in base ad accordi internazionali. L'unico aspetto positivo è stato la celerità dei soccorsi e questo può essere anche utilmente sottolineato. Non credo, però, che sia opportuno aprire un dibattito, prendendo spunto da questo fatto, o sulla stampa, o nelle Aule parlamentari, per sostenere che le esercitazioni nel nostro Paese non debbano essere fatte e per dire che che rinunciamo, ancora una volta, alla nostra sovranità; oppure - come surrettiziamente si tende ad affermare - che non ci debbano neppure essere le Forze armate.

adoperarci perché esistano le condizioni affinché la pace possa effettivamente realizzarsi, è altrettanto ovvio che le esercitazioni debbano svolgersi con maggiori misure e attenzioni per la sicurezza della popolazione.

La storia del secolo scorso ci dice che l'Europa deve grande riconoscenza alla nazione americana perché, per almeno due volte, è intervenuta con largo dispendio, non solo di mezzi, ma di vite umane, per difendere

Signor Presidente, volevo preventivamente ricordare che l'intervento della senatrice Pisa, come il mio, sono fatti a nome dei Gruppi della Sinistra di questo Parlamento, che insieme vogliono esprimere un sincero cordoglio alle famiglie dei militari statunitensi colpiti dalla sciagura, alle famiglie dei feriti, ai quali auguriamo auguriamo di cuore l'immediata guarigione, e alle famiglie di coloro che sono morti. Non possiamo però, accanto a questo cordoglio, non porci alcune domande, non fare alcune riflessioni che questo incidente chiama in causa,

soccorsi. La nostra preoccupazione è grande per il pericolo che i voli militari rappresentano sui cieli del Veneto. Siamo molto preoccupati, come diceva la senatrice Pisa, per l'addestramento dei soldati USA sul greto del fiume

Su Vicenza non possiamo non soffermarci un attimo, nel momento in cui si sta pensando di costruire una nuova base militare a 1.500 metri dal centro della città, dalla basilica Palladiana. Cosa potrebbe accadere se un simile incidente avvenisse sui cieli

come in questo caso in cui ci viene addirittura richiesta la rinuncia alla giurisdizione. Il commissario straordinario Costa, delegato dal Governo ad occuparsi di questo, continua a dire che il suo compito è esattamente di garantire «il minore impatto possibile sulla popolazione della costruzione della nuova base». Chiedo davvero al commissario Costa se può escludere che un incidente simile possa verificarsi in avvenire sui cieli di Vicenza. La caduta di questo elicottero ha spaventato veramente la popolazione di Vicenza. Quali compensazioni il commissario può garantire alla popolazione vicentina? La tragedia di oggi, ancora una volta, ha confermato i timori dei cittadini che anche in questi giorni stanno bloccando la bonifica dell'aeroporto Dal Molin, funzionale alla realizzazione della nuova base

di far rispettare - e stavolta possiamo parlare a ragion veduta di sicurezza - la sicurezza dei nostri cieli, del nostro Paese. Chiedo anche al Governo che fine ha fatto l'ordine del giorno approvato da quest'Aula nel mese di febbraio e nel quale si impegnava il Governo a indire la Seconda conferenza nazionale sulle servitù militari, all'interno della quale ridiscutere la presenza delle basi militari italiane NATO e di potenze straniere nel nostro territorio. fino alla convocazione di quella conferenza, prevista peraltro dal programma dell'Unione, vi fosse una moratoria nella costruzione della base. Oggi riaffermiamo queste richieste perché pensiamo che in tempo di pace i nostri cieli e i nostri territori non possano continuare ad essere teatro di esercitazioni e

Vorrei esprimere, a nome di Alleanza Nazionale, agli Stati Uniti, alle Forze armate americane, a coloro che operano nella base di Aviano,

Purtroppo aveva ragione il collega Stracquadanio: ad un certo punto, qualcuno ha approfittato ancora una volta di una disgrazia

del dilettantismo politico, dimostrando irresponsabilità. Stiamo vivendo in un paradosso: abbiamo di fronte tre interventi di chi fa parte del Governo, i quali si rammaricano della presenza americana, del fatto che non siano stati rispettati i programmi, della necessità di ridurre la presenza e poi, bellamente, rimangono nel Governo, facendo così i dilettanti. Si divertono a scagliare frecce ma poi rimangono in un Governo che, purtroppo, gli italiani hanno nominato e di cui debbono rendersi conto, il quale naturalmente, per forza, rispetta i patti internazionali, gli accordi ed ha un atteggiamento quanto meno responsabile. Da questa parte si difende l'operato, si ricorda la gratitudine che il nostro Paese deve avere nei confronti degli Stati Uniti; dall'altra parte, coloro che per quarant'anni si sono etichettati come comunisti e sognatori del socialismo reale si dimenticano che, se non avessimo avuto gli americani, dai piani emersi dalle forze del Patto di Varsavia, è emerso chiarissimamente che erano che erano pronti ad attaccarci, non appena vi fosse stato un minimo di debolezza o se non avessimo avuto la capacità della deterrenza dell'ordigno nucleare. Non si vergognano di affermare, di chiamare disturbo la presenza degli americani. Non si vergognano di questa ingratitudine. Ma avrei voluto vedere - la collega Pisa se ne è andata - in quali condizioni avreste vissuto se aveste fatto parte di quella congerie di satelliti, rovinata dal comunismo; se aveste fatto parte di quelle popolazioni che hanno perduto milioni di persone per la ferocia di questo sistema politico. Adesso, belli belli, mi venite a dire che gli americani disturbano e che è il caso di ridiscutere la loro presenza. Non avrei raccolto queste meschinità se non fosse necessario lasciare agli atti

ringrazio il Sottosegretario per le informazioni che ci ha dato. Poteva limitarsi a questo ringraziamento l'intervento che faccio a nome del Gruppo Forza Italia,

Esprimiamo, dunque, il nostro cordoglio, la nostra simpatia per le truppe americane che si trovano in Italia a difesa della nostra sicurezza. Ma vedo che il Governo ha delle difficoltà a far passare questo stato, questa condizione, questa necessità in cui si trova il nostro Paese di essere garantito da quelle Forze armate che ci hanno dato la libertà (lo ha detto molto bene il senatore Ramponi poco fa), mentre secondo l'Unione Sovietica, verso la quale ci si rivolgeva un tempo, e mi pare che con accenti ideologici non siamo molto lontani da quella concezione, le Forze armate servivano a Praga ed a Budapest per schiacciare i vagiti di libertà che si manifestavano in quei Paesi. Siamo quindi grati agli Stati Uniti d'America, perché si trovano oggi nel nostro Paese a difenderci contro un'altra forma di grave pericolo,

lo ha detto con precisione) da quella che era una programmata aggressione del nostro sistema politico e quindi della nostra area geografica. non avrei fatto questo discorso e mi sarei limitato ad esprimere il cordoglio alla Nazione americana se non avessi sentito nelle dichiarazioni delle senatrici dell'estrema sinistra gli echi di coloro che nelle piazze d'Italia hanno, non molto tempo fa, gridato: «Fuori l'Italia dalla NATO, fuori la NATO dall'Italia». No, noi riteniamo che la dimostrazione e il sacrificio di questi militari siano un esercizio assolutamente legittimo. Mi spiace di dover

di me parlerà il senatore Zanone. Spero che da lui vengano più rassicuranti notizie circa il fatto che questa rappresenta nell'area della maggioranza soltanto un'eccezione malaugurata, secondo me,

diversi da quelli ideologici e forse anche in questo una concezione ideologica c'è. Per tali ragioni, la nostra riconoscenza, la nostra vigilanza, il nostro supporto agli Stati Uniti d'America e alle loro Forze armate restano

il Gruppo dell'Ulivo esprime la propria partecipazione, associandosi in ciò a quanto ha dichiarato il rappresentante del Governo, al lutto delle famiglie dei militari americani caduti in un'operazione di addestramento, ed esprime solidale cordoglio al Governo americano e alle sue Forze armate, cui l'Italia è legata da un rapporto di alleanza, sulle cui rassicurazioni, senatore Selva, non occorre dare attestati in questa sede. L'attestato viene dalla storia del secondo Novecento, del rapporto fra l'Italia e l'America nel quadro della solidarietà atlantica ed oggi del partenariato fra

e ad evolversi, nel nuovo concetto strategico ormai allo studio da otto anni da parte dei Governi ed in sede di Assemblea parlamentare della NATO.

nel funzionamento dei grandi sistemi militari, richiedono in questa sede una duplice avvertenza. In primo luogo, sono momenti in cui il vincolo dell'alleanza si mostra con più chiarezza, perché la solidarietà diventa un fattore anche politicamente importante proprio nei momenti della sfortuna e della disgrazia. Al tempo stesso, credo che le ore della sfortuna siano le meno idonee a porre argomenti di confrontazione che sono viceversa più che legittimi in altra sede e in altri momenti della discussione. Sulla presenza delle basi americane in Italia; sulla ridefinizione del sistema delle servitù militari, che com'è noto è oggetto di ampia indagine da parte alla Commissione difesa alla Camera dei deputati; e in particolare sulla nuova infrastruttura di Vicenza, anche il Senato non ha mancato di apprezzare diversi punti di vista e non mancherà di continuare a farlo, avvalendosi degli impegni di informazione e di concertazione che sono stati presi in questa sede dal Governo. Le senatrici Pisa, Rubinato e Valpiana hanno posto hanno posto poc'anzi, in questa nostra breve sessione, un problema di grande delicatezza e complessità quale è quello della riserva di giurisdizione. Certamente, l'importanza del tema credo non sfugga a nessuno e forse meriterebbe di essere esaminata anch'essa in una luce nuova nel quadro della politica europea di sicurezza e di difesa, che è il nuovo quadro di riferimento delle nostre relazioni internazionali in materia militare; un quadro di riferimento di cui - credo che

Vorrei solo osservare, se lei me lo consente signor Presidente, che la questione della giurisdizione non manca nemmeno di precedenti, perché fu fatta valere seppure con un quadro diverso, per esempio, dal Governo italiano